la seduta di oggi si concluderà alle ore 18 con la votazione della questione pregiudiziale sul disegno di legge concernente l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario. I tempi della discussione della questione pregiudiziale non sono conteggiati nella ripartizione dei tempi assegnati ai Gruppi. Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

i tempi doverosi per un dibattito esaustivo su un argomento complesso come questo. Il perno della mia relazione, seppur sintetica, verterà sulle modifiche apportate al testo originario,

e abbia la finalità di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio; altresì, sono richiamati i principi solidaristici di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione. Lo stesso principio viene ribadito nel successivo articolo 2, che prevede una vera e propria clausola di limitazione delle intese da parte del Presidente del Consiglio, al fine di assicurare la coesione nazionale e di tutelare l'unità giuridica ed economica, nonché l'indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie. È previsto che il Presidente del Consiglio, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, possa limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione nell'atto di iniziativa. Come detto, il lavoro in Commissione ha portato addirittura ad inserire nuovi articoli e a sostituirne altri. È il caso per esempio dell'articolo 3, che è stato completamente riscritto

Esso prevede inoltre che i decreti siano adottati solo dopo l'entrata in vigore delle norme che stanziano le relative risorse finanziarie. Sono state previste anche norme sulla perequazione. L'articolo 4 ci ricorda che i LEP devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, per evitare disparità di trattamento tra le Regioni: è bene ricordare che, laddove dalla loro determinazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, detto trasferimento è autorizzato solo in seguito all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie, coerenti con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio, con riferimento all'intero territorio nazionale, al fine di evitare disparità di trattamento tra le Regioni. Norme metodologiche sono contenute nell'articolo 5, che disciplina le modalità dell'intesa, e nell'articolo 6, che invece disciplina il trasferimento delle funzioni dalle Regioni agli enti locali. L'articolo 7 invece

garanzie dei LEP, può intervenire per farle cessare o parzialmente ridurre. Per effetto della novella apportata all'articolo 7 in ogni caso, lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. L'articolo 8 è invece relativo alla commissione paritetica di valutazione degli oneri derivanti dalla delega di funzioni, che viene data alle Regioni. L'articolo 9 stabilisce invece un principio che riprende l'articolo 1, che riguarda la coesione e l'unità nazionale, stabilendo che le intese non possono pregiudicare l'entità delle risorse da attribuire alle altre Regioni ed è garantita la perequazione fiscale per i territori con minore capacità fiscale e per l'insularità. L'articolo 10 è una norma di garanzia sempre a vantaggio dell'unità nazionale e della coesione sociale, anche al fine di eliminare *deficit* infrastrutturali tra le diverse aree, unificando diverse fonti di finanziamento statale e in conto capitale anche per le Regioni che non concludano le intese. L'articolo 11, infine, è una norma che reca precetti transitori e che stabilisce il prosieguo delle proposte d'intesa che abbiano avuto inizio per le Regioni che le abbiano già richieste, disponendo altresì che il predetto provvedimento di legge si applichi anche alle Regioni a Statuto speciale.

il collega Della Porta ha spiegato compiutamente i dieci articoli del disegno di legge il significato di ogni singola parte che compone questo importante provvedimento che, finalmente, è approdato nell'Aula del Senato dopo un lungo *iter* in Commissione affari costituzionali, durato otto mesi (dal 23 marzo a fine novembre), con 58 soggetti auditi, 66 documenti acquisiti, 70 sedute di Commissione, 649 emendamenti, 401 votazioni effettuate, comprese quelle degli ordini del giorno, 84 emendamenti approvati (un numero cospicuo), di cui 44 delle opposizioni, e 51 ore complessive dedicate all'esame del testo. Tutto si può dire, ma non che il presidente Balboni, tutta la Commissione, la maggioranza e il Governo non abbiano consentito un ampio dibattito in Commissione affinché

5, che voglio ricordare a tutti perché tutti noi siamo chiamati a rispondere al dettato costituzionale e ad esserne interpreti, come legislatori.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

di una Costituzione in cui tutti ci riconosciamo e che deve trovare finalmente attuazione. Il rispetto della Costituzione implica anche l'attuazione della riforma del Titolo V, è stato approvato nel 2001 e portato avanti da un Governo e da una maggioranza di centrosinistra ed ha avuto

*referendum* sulla *devolution* portato avanti dal centrodestra e il *referendum* di Renzi sulla modifica della Costituzione, hanno avuto parere negativo dal corpo elettorale.

si è espresso anche in altre occasioni attraverso, due *referendum*: uno si è tenuto in Lombardia e uno in Veneto, il 22 ottobre del 2017, che ha sancito che la maggioranza dei cittadini di quei territori, su iniziativa dei rispettivi Presidenti e delle rispettive Giunte, aderiva all'idea di concedere maggiore autonomia alle proprie Regioni, proprio nel rispetto pieno della Costituzione e del Titolo V.

Anche questo è un elemento fondamentale: il rispetto della volontà popolare. Non ci fermiamo qui, però, perché anche la Regione Emilia-Romagna, in prima istanza, e poi quasi tutte le altre Regioni a statuto ordinario hanno aderito al percorso dell'autonomia differenziata. Delle quindici Regioni a statuto ordinario solo l'Abruzzo non ha chiesto, nel corso della scorsa legislatura, forme aggiuntive di autonomia. quindi evidente che ci sono una volontà e una spinta da parte dei territori a ottenere questo riconoscimento e il Parlamento aveva il dovere di delineare un percorso perché queste richieste, nel pieno rispetto della Costituzione, potessero trovare attuazione.

di una scelta volta a rendere l'attuazione dell'autonomia più condivisa e più trasparente possibile, con il coinvolgimento più ampio degli enti territoriali e del Parlamento. Come relatori, quindi, non possiamo che rigettare al mittente l'accusa di taluni che ritengono questo percorso incostituzionale. Ricordiamo che un'altra delle richieste della scorsa legislatura, presentata da alcune forze politiche, era quella di subordinare il riconoscimento dell'autonomia differenziata alla definizione dei LEP e all'eventuale finanziamento, qualora si rendesse necessario, non solo per quelle che chiedessero l'autonomia differenziata, ma per tutte le Regioni. Ebbene, tale requisito è contenuto in questo disegno di legge, in questo disegno di legge, nel quale è stato previsto anche il riconoscimento del fondo perequativo per i territori maggiormente in difficoltà.

Il fatto che l'autonomia possa essere riconosciuta anche per ambito di materia non implica necessariamente che l'intera materia possa essere chiesta o attribuita, anche solo parziale. Quindi non ravvisiamo pericoli per la coesione e l'unità nazionale, anche perché comunque l'ultima parola, a fronte della richiesta di una singola Regione, spetterà in prima istanza al Governo, ma in istanza finale al Parlamento sovrano, rappresentante della volontà dei cittadini, che dovrà esprimersi a maggioranza assoluta. quindi, non c'è nulla da temere e questo disegno di legge quadro è un punto di equilibrio che riteniamo si sia raggiunto all'interno della Commissione tra le varie istanze delle forze di maggioranza, ma anche di concerto con alcune posizioni delle opposizioni e dispiace che stia prevalendo una contrarietà di natura politica, rispetto a una contrarietà di merito, che onestamente non comprendiamo. Attraverso questa riforma vorremmo, una volta per tutte, chiarire un concetto: l'autonomia è un'opportunità per tutti i territori, per tutte le comunità e per tutte le Regioni. Non è la rivendicazione di un territorio o di un'area geografica a discapito di un'altra, rappresenta semplicemente un percorso attraverso il quale le competenze e le risorse che oggi sono gestite dallo Stato centrale possono

concedendo libertà di manovra ai territori che hanno specificità sociali ed economiche che meritano meccanismi di governo del territorio fondati sul principio dell'autonomia. Questo è l'intento della battaglia autonomista nel suo complesso, ma anche di questo disegno di legge. Noi respingiamo al mittente l'accusa che questa riforma spacchi il Paese e che rappresenti un favore al Nord a discapito del Sud. È un'opportunità per tutti, come ho detto, e una scommessa per quei territori che potrebbero usare meglio la gestione di risorse e servizi rispetto allo Stato centrale. Riteniamo quindi che questa sia un'occasione storica per dare finalmente concreta attuazione alla Costituzione, al Titolo V e agli articoli 116 e 119, con la definizione dei LEP. È una grande opportunità e un riconoscimento per tutti coloro che hanno lottato in questi anni per far vincere la cultura autonomista rispetto a quella centralista che, lo voglio ricordare, non ha funzionato e non ha risolto i problemi e i divari territoriali, che oggi esistono perché c'è uno Stato centralista. Noi siamo convinti che, attraverso questa riforma,

molte delle gravi criticità che sono state evidenziate da più parti nel corso degli ultimi mesi. In particolare, rimangono intatti i profili di incostituzionalità per un'evidente contrasto con numerose disposizioni costituzionali, cioè gli articoli 1, 3, 4, 33, 34, 53, 70, 116, 117 e 119. Voglio dire, Presidente, in via preliminare, che non è l'autonomia in sé ad essere contro la Costituzione, ma la sua declinazione come autonomia differenziata, che spacca definitivamente il Paese, aumenta i divari territoriali e fa crescere le diseguaglianze sociali. L'autonomia sancita fra i principi fondamentali della Costituzione, all'articolo 5, era stata immaginata in totale connessione con i principi della democrazia, della solidarietà, dell'uguaglianza e della sovranità popolare. È impregnata di questi principi e il riferimento all'unità, anch'esso contenuto nell'articolo 5, inscrive l'autonomia in un orizzonte costruito attorno ai diritti e attorno all'emancipazione. Non è contro, ma è parte dell'unità nazionale: tutto il contrario, Presidente, della secessione dei ricchi che voi state facendo con questo disegno di legge, in totale contrasto col progetto costituzionale di uguaglianza sostanziale, così come sancito dall'articolo 3 della Carta. Questa riforma produrrà la cristallizzazione delle differenze esistenti fra i territori e consentirà alle Regioni più ricche di trattenere risorse per garantire i propri cittadini, mentre i territori più fragili, il Mezzogiorno innanzitutto, ma anche le aree più periferiche e più interne, avranno difficoltà insormontabili a raggiungere i livelli di sviluppo e di benessere sociale che servirebbero. Non bastavano, evidentemente, né il taglio del fondo perequativo e nemmeno il taglio da 7,6 miliardi alle risorse del PNRR destinate al Sud. Con questo disegno di legge date il colpo di grazia definitivo a tutta quella parte del Paese dov'è più acuta la sofferenza sociale. I divari territoriali diventano potenzialmente irreversibili, con il rischio evidente di tensioni che mettono a rischio l'unità nazionale così come l'abbiamo conosciuta. Con questo disegno di legge scompare il regionalismo solidale disegnato dalla nostra Costituzione, quell'idea di autonomia che che immagina il territorio come spazio di riconoscimento della dignità sociale, che si inserisce - quella sì, armonicamente - nel progetto di costruzione dello Stato sociale. La vostra idea, che è tutta dentro questo disegno di legge, si fonda su un regionalismo non più solidale, ma competitivo e rappresenta una rottura con il principio di uguaglianza. È un progetto che nasce da lontano, come sappiamo, e che accentua le criticità contenute nella riforma del Titolo V del 2001, riforma già profondamente sbagliata, che avrebbe necessitato, anche alla luce dell'esperienza degli ultimi anni, di una profonda revisione, come viene fatto peraltro dal disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare per il quale sono state recentemente raccolte 100.000 firme e che, per una questione logica, oltre che regolamentare, quest'Assemblea avrebbe dovuto affrontare prima di legge Calderoli e non dopo, come invece faremo. Il vostro progetto, anziché correggere le distorsioni della riforma del 2001, ne rende ancora più gravi gli effetti e la stessa circostanza che l'autonomia differenziata sia un processo ineludibile, perché previsto dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione, non esonera gli attori politici dal rispetto dei principi costituzionali fondamentali cui tutte le cui tutte le norme giuridiche debbono conformarsi, comprese le leggi di revisione costituzionale. Questo significa che lo stesso principio di differenziazione andrebbe declinato nel principio costituzionale dell'eguaglianza sostanziale, per il quale occorre trattare in modo uguale situazioni eguali e in modo differente situazioni differenti, facendo del trattamento differenziato la chiave di volta del principio di non discriminazione e del principio pluralistico. Il principio di differenziazione stesso, già contemplato prima della riforma del 2001, non è infatti di esclusiva portata dell'articolo 116 della Costituzione, ma trova un riferimento specifico anche nell'articolo 117 che, nel terzo comma, assegna una serie di materie alla potestà legislativa concorrente di ciascuna Regione, il che evidentemente già implica in quelle materie la possibilità di una differenziazione Regione per Regione, come gli articoli 118 e 119, che attengono ai profili amministrativi e finanziari del principio di autonomia costituzionale. Il testo che oggi la Commissione propone all'Assemblea tradisce lo spirito della Costituzione con una torsione pericolosa e inaccettabile e contrasta inoltre con gli articoli 70 e seguenti, perché svuota di potere il Parlamento nelle sue prerogative legislative, non essendo sufficienti le timide modifiche apportate in Commissione, che hanno soltanto smussato alcuni aspetti senza però cambiarne la sostanza. Un decreto legislativo, peraltro, come tutti sappiamo, è cosa ben differente da una legge ordinaria. Ancora, sul tema delle risorse economiche, il criterio della spesa storica vale in riferimento alla sentenza n. 275 del 2016 della Corte sulla necessità cioè che sia lo Stato con il suo bilancio a soddisfare i diritti inviolabili dei cittadini, qualunque sia il territorio in cui vivono. Peraltro, in riferimento alla spesa come criterio di ripartizione delle risorse, esso denuncia e conferma le profonde differenze già esistenti, rendendo evidente la palese illegittimità del criterio prospettato, senza dimenticare la disposizione degli articoli 2 e 53 della Costituzione, secondo i quali la solidarietà economica e tributaria opera a livello nazionale e non regionale. Infine, un'ultima notazione in materia di istruzione. Questo testo, dal nostro punto di vista, è in palese contrasto con gli articoli 33 e 34 della Costituzione, che assegnano alla scuola un compito decisivo su cui si fonda la convivenza democratica del Paese, cioè l'idea secondo la quale la costruzione della cittadinanza, la condivisione di valori e il senso di appartenenza si debbano determinare mediante un'offerta formativa omogenea, in grado di assicurare la sostanziale parità di trattamento tra coloro che fruiscono dell'istruzione: anche questo, drammaticamente, viene messo in discussione. Per tutte queste ragioni, vi chiediamo di fermarvi e, a tal fine, abbiamo presentato, oggi più che mai, una pregiudiziale di costituzionalità. dell'Istituto d'istruzione superiore «Giovan Battista Odierna» di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento.

Signor Presidente, siamo chiamati ad approfondire e legiferare attorno a un tema come quello dell'autonomia differenziata che per molti versi ha rappresentato una bandiera ideologica, con la quale un pezzo dell'attuale maggioranza ha costruito le sue ragioni e in qualche caso anche le sue fortune politiche. Non vi è dubbio che dietro a questa impostazione, che oggi viene portata all'attenzione dell'Assemblea, vi sia un patto leonino all'interno di questa maggioranza, sulla base del quale cioè l'autonomia differenziata debba procedere come pegno da pagarsi al partito del vice *premier* Matteo Salvini, la Lega-Salvini Premier, ex Lega Nord, in cambio dell'*affidavit* a un altro pezzo di maggioranza,

In mezzo, non si capisce bene quale sia la posizione di Forza Italia e del residuo di moderatismo e riformismo connesso all'interno della coalizione di Governo, ma tant'è: è questa la stagione che siamo chiamati a vivere. Dentro questa compressione, dentro questo patto leonino, emerge un testo che inevitabilmente porta con sé - sia questo che quello che poi affronteremo sul premierato - il marchio di fabbrica del pasticcio. Anche su questo occorrerebbe intendersi, e lo dico in particolare al ministro Calderoli qui presente. La forza politica che noi qui oggi rappresentiamo non si ispira alla logica del sindacalismo territoriale. riteniamo che si debba affrontare un tema così delicato evitando di contrapporre a una dinamica quasi ideologica, che è stata utilizzata in questi anni come una clava per far fronte ai bisogni e alle esigenze di un pezzo di territorio, una logica contrapposta e specularmente Insomma, per dirla con una battuta: non possiamo assistere ad un dibattito tra fautori di una Lega Nord e fautori di una Lega Sud, perché questo spaccherebbe intimamente il Paese e porterebbe a perdere di vista vista la dimensione reale della riorganizzazione statuale. Il tema non è rivendicare competenze partendo da una logica di sindacalismo territoriale. Il tema è come inserire la questione delle autonomie all'interno del presupposto fondamentale sancito dall'articolo 5 della nostra Costituzione, che non a caso De Gasperi definì essere il cuore della nostra Carta costituzionale, secondo cui la Repubblica, una e indivisibile, uniforma il proprio ordinamento sulla base delle autonomie che vengono riconosciute come preesistenti. Se è questo lo spirito con il quale occorre approcciarsi, è evidente che bisogna sollevare le incongruenze dal punto di vista costituzionale,

legge all'ordine del giorno cozza in maniera clamorosa con l'articolo 3 della Costituzione, che sancisce il principio di eguaglianza dei cittadini come elemento strutturale dell'identità repubblicana.

né tantomeno di come finanziarli, perché evidentemente, non avendoli definiti, figuriamoci se possiamo dire come li finanziamo. È una sorta di *affidavit,* è una cambiale in bianco, è qualcosa che viene rimesso al futuro, in una dimensione generica nella quale la buona volontà e le speranze sostituiscono la legge. È di tutta evidenza che in un Parlamento liberale non si può sostituire la buona volontà a un sistema di leggi e di garanzie.

volontariamente il condizionale, perché poi cercheremo di capire come arriverà in fondo; di certo, infatti, vi servirà per fare un po' di campagna elettorale per le prossime elezioni europee, ma poi vedremo anche quanto servirà dal punto di vista della raccolta del consenso raccontare queste favole. Il tema vero è che, se questo disegno di legge arrivasse fino in fondo, avremmo tre livelli di ordinamento regionale: avremmo le Regioni a statuto ordinario, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome (anzi quattro a questo punto) e poi le Regioni differenziate. È di tutta evidenza che tutto questo barocco ordinamento cozza contro l'articolo 97 della Costituzione, che sancisce il principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Per le materie portate all'interno dell'articolo 117,

dovremmo fare il mercato europeo dell'energia siamo qui a discutere se il Molise o la Basilicata possano gestire in maniera autonoma ed esclusiva una materia così delicata. Già questo la direbbe lunga rispetto al fatto che non si persegue il buon andamento della pubblica amministrazione. Ma mettetevi nei panni di un imprenditore che ha diverse strutture sul nostro territorio nazionale e, per fare lo stesso investimento, in una Regione deve chiedere un certo tipo di autorizzazioni, in un'altra un altro tipo e mentre in una riceve una risposta positiva, nell'altra ne riceve una negativa.

compongono l'esigenza di suggellare la insostenibilità costituzionale di questo provvedimento. Il primo è che qui non si parla di sussidiarietà, e lo dico in particolare agli amici di Forza Italia, con cui abbiamo molte molte volte preso diverse posizioni in questa direzione. Qui si parla di centralismo regionale: non si dà nessuno spazio, nessuna garanzia, nessuna previsione al ruolo degli enti locali, Comuni, Province e Città metropolitane, che non sono sottordinati, ma sono equiordinati rispetto all'articolo 114 della Costituzione. E addirittura, leggendo l'articolo 118, si vede che il principio di sussidiarietà parte dai Comuni e invece voi, dentro questa dimensione di creazione di un meccanismo di centralismo regionale che vuole sostituirsi allo Stato, non prevedete in alcun modo un meccanismo automatico di devoluzione verso il sistema delle autonomie. Questo viene affidato alla buona volontà dei cosiddetti governatori, che evidentemente

perché l'articolo 70 della Costituzione viene sostanzialmente messo tra parentesi. Saremo chiamati a votare un'intesa tra lo Stato e le Regioni come se fosse un'intesa tra la Repubblica italiana e uno Stato estero, che poi sarà inemendabile da questa Assemblea. Pertanto, dovremo prendere per buone tutte le decisioni e non avremo più nessuna possibilità di entrare nel merito. Ma vi pare che sia possibile costruire realmente un sistema articolato di autonomia oppure ci si sta avviando verso una grande confusione? Questa è la nostra estrema preoccupazione per la quale chiediamo di fermarci e, se vogliamo realizzare l'autonomia differenziata, facciamolo sul serio e non come manifesto elettorale destinato a perdersi molto presto.

*(M5S)*. Signor Presidente, devo esprimere preliminarmente la mia costernazione da senatore della Repubblica nel constatare che

sommato, in pochi minuti di dibattito, come se fosse un provvedimento di concessione di una minuscola contribuzione finanziaria a qualche sagra di paese. È assolutamente inaccettabile questo metodo, che offende l'istituzione parlamentare e ridonda, purtroppo, nella disaffezione della gente nei confronti della politica e purtroppo nei confronti del Parlamento. Passo poi al merito delle questioni da affrontare sotto il profilo della pregiudiziale di costituzionalità. Questo provvedimento rassegna almeno dieci aspetti di incostituzionalità. Sappiamo tutti che ne basta uno perché cada sotto la falce della Corte costituzionale. Questo ne ha ad esuberanza, ne ha una decina, e forse anche una dozzina. Il tempo che ho a disposizione purtroppo è limitatissimo e, quindi, farò una carrellata molto veloce. Innanzitutto questo provvedimento modifica in profondità l'assetto costituzionale attraverso un procedimento anomalo, quello della legge ordinaria, disapplicando l'articolo 138 della Costituzione, che istituisce un procedimento aggravato. Basta già questo per consegnare il provvedimento nelle mani della Corte costituzionale per la falcidia dello stesso. viene modificato l'articolo 116, comma primo, che prevede categorie differenziate (Regioni a Statuto speciale e Regioni a statuto ordinario). Se tutte le Regioni a statuto ordinario optano per il regionalismo autonomo differenziato, cade la differenza categoriale viene modificato di fatto l'articolo 116, ma non attraverso il procedimento tipico dell'articolo 138. l'articolo 117 istituisce la categoria della competenza concorrente dello Stato. Se questa competenza viene espropriata allo Stato e dislocata presso le Regioni, abbiamo un'altra modifica del testo costituzionale. Cessando la competenza concorrente, si modifica l'articolo 117, e lo si modifica con legge ordinaria. Questo è un altro motivo di incostituzionalità. Continuo rapidamente. La cosa più aberrante è avere legato la fruizione dei diritti sociali e civili, garantiti dalla Costituzione

che viene a sostituire lo *ius civitatis*. Cioè, se io appartengo a un determinato territorio, avrò pienezza di fruibilità di questi diritti; se non appartengo a quel territorio, purtroppo rimango circuitato. Questo segna una violazione immancabile e innegabile dell'articolo 119, oltre che dell'articolo 3 della Costituzione. Ancora, un'altra violazione della Costituzione, perché non è stato seguito il metodo dell'articolo 138, è in relazione all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Cosa dice il Trattato? L'Unione mira a ridurre il divario nei livelli di sviluppo delle varie Regioni

l'articolo 174 del Trattato, violiamo l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, che sancisce la priorità e la inderogabilità dei principi dell'ordinamento comunitario da parte della legge interna.

veramente il fulcro dell'incostituzionalità di questa riforma nel seguente passaggio argomentativo. Esiste un principio, asseverato da copiosa e consolidata giurisprudenza costituzionale, che dice che il principio di ragionevolezza, inteso come principio di non contraddizione e di coerenza, è immanente all'esercizio del potere legislativo e segna un limite invalicabile alla cosiddetta onnipotenza del legislatore. Qui abbiamo posto in essere un disegno di legge che è illogico *(Applausi)* e viola il principio di ragionevolezza immanente al procedimento legislativo. Ciò lo dice autenticamente l'articolo 4, comma 1, ricordato dal relatore, quando stabilisce che la condizione perché venga attuata in concreto la devoluzione

L'articolo 1346 del codice civile enuclea il principio che, quando un atto, un provvedimento, un negozio è sottoposto a condizioni impossibili, è radicalmente nullo.

È una legge irrealizzabile e, se realizzata, sarà con ogni probabilità cancellata dalla Corte costituzionale.

1947 in Assemblea costituente Pietro Nenni, discutendo del federalismo regionale, che, in una Nazione dove all'antagonismo sociale tra poveri e ricchi si unisce il dislivello tra le Regioni settentrionali e quelle meridionali,

Quali riforme socio-economiche voi avete fatto per creare il terreno favorevole alla riforma autonomistica? Quella di aver svuotato il fondo perequativo infrastrutturale di 4,7 miliardi. Nello 4,7 miliardi. Nello stesso ristretto arco temporale avete azzerato il fondo perequativo e volete realizzare l'autonomia differenziata. È una cosa di cui sinceramente vi dovreste vergognare.

Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, noi ci troviamo di fronte a un'operazione elettoralistica consumata sulla pelle dei cittadini italiani e - voglio dirlo subito - sulla pelle di tutti i cittadini italiani, di tutte le parti del nostro Paese. Non è vero, come qualcuno sostiene, anche tra coloro che sono critici del provvedimento governativo sull'autonomia differenziata, che soltanto le popolazioni del Mezzogiorno correrebbero rischi. Da questo disegno di legge sbagliato, divisivo, pericoloso, trarranno grossi danni, in caso di sua attuazione, tutti i cittadini di questo Paese, tutte le Regioni di questo Paese, quelle più avanzate, quelle economicamente meno avanzate e, in generale, il sistema istituzionale italiano. *(Applausi)*. Noi avremo modo, nel corso della discussione generale e nelle dichiarazioni di voto che si alterneranno, di spiegare come mai vada contrastato questo pericoloso disegno di suddivisione della popolazione italiana in cittadini di serie A e di serie B e di suddivisione del sistema delle Regioni italiane in Regioni di serie A e di serie B. questione pregiudiziale, e quindi di richiesta di non passare all'esame del provvedimento, io ritengo necessario mettere l'accento su alcune questioni questioni di metodo e di sostanza, che configurano un contrasto palese tra il modo in cui il Governo ha scelto di procedere e i principi e le norme della nostra Costituzione. La prima questione su cui dobbiamo tutti riflettere è quella che consegue alla scelta di rendere possibile, come prevede il disegno di legge governativo, il trasferimento non soltanto di alcune funzioni e di alcuni ambiti di materie alle Regioni che ne fanno richiesta, ma anche il trasferimento di interi ambiti di materie. In questo modo, compiremmo un'operazione per la quale l'attuazione del comma 3 dell'articolo 116, che prevede la possibilità di conferire ulteriori margini e condizioni di autonomia ad alcune Regioni, diventa praticamente una norma dissolutoria del comma 1 di quell'articolo, che concede uno statuto particolare alle Regioni a Statuto speciale, che proprio così vengono chiamate. Verremmo così a perdere una distinzione fondamentale del nostro ordinamento. E questo è un elemento che sembra tecnico, ma è eminentemente politico, perché comunica il tasso di confusione con cui l'operazione è stata portata avanti e gli effetti disgregativi che essa può produrre. Vi è un altro elemento su cui io credo che dobbiamo mettere l'accento, perché ha molto in comune anche con altre iniziative di rango costituzionale che la maggioranza sta portando avanti. Mi riferisco al disegno di legge sul premierato, sul quale è in corso la discussione generale in Commissione. Un altro elemento molto critico è quello della decisione palese, chiara, di mortificare il Parlamento nell'attuazione dei procedimenti di conferimento di ulteriori margini di autonomia alle Regioni che ne faranno richiesta. La mortificazione del Parlamento è totale

causare un danno molto grande, all'interno del nostro sistema istituzionale, con una legge - quella che stiamo esaminando - che è ordinaria. una legge di rango inferiore a quello che avrà la legge di approvazione dell'intesa, che arriverà al nostro esame se noi non riuscissimo - come io mi auguro - a fermare questa operazione. La legge di approvazione dell'intesa sarebbe una legge che richiede la maggioranza assoluta

La nostra opinione, che abbiamo sostenuta inutilmente in Commissione, è che questa procedura doveva iniziare con una legge costituzionale. La cornice doveva essere una legge costituzionale e, dentro la legge costituzionale, doveva trovar sede l'eventuale legge di approvazione dell'intesa, da approvarsi a maggioranza assoluta in Parlamento. non è il solo atto di violenza che si consuma verso il Parlamento. C'è n'è un altro, molto grave, e cioè il fatto che al Parlamento è negata qualsiasi possibilità di emendare il testo dell'intesa eventualmente raggiunta tra Esecutivo nazionale ed Esecutivi regionali. C'è un disprezzo verso i corpi legislativi che si estende dal Parlamento nazionale ai consigli regionali stessi, quindi alle Assemblee legislative regionali. I corpi legislativi non possono mettere bocca in questa procedura: possono soltanto dire in blocco sì o no, e capite che questo non va assolutamente bene. Secondo me, configura un profilo profilo di illegittimità piuttosto chiaro che ci sarà modo e maniera di mettere in evidenza se, appunto, la battaglia parlamentare nel Paese che abbiamo intenzione di fare contro questo provvedimento non raggiungesse gli esiti che speriamo. Ma c'è di più: io considero un atteggiamento anti-istituzionale e palesemente in contrasto anche con la necessità di leale collaborazione tra tutti i livelli dello Stato il modo in cui si è andati avanti, senza cercare l'unanimità nella Conferenza delle Regioni, diversamente da quanto altri Governi che si erano cimentati in questo compito avevano provato a fare, disegnando il percorso dell'autonomia differenziata. La Conferenza delle Regioni è stata scientemente spaccata, non si è cercata un'intesa e - come abbiamo purtroppo inutilmente sottolineato in più occasioni durante il dibattito in Commissione - totale è il mancato coinvolgimento degli enti locali, Comuni e Province. Attenzione: noi non possiamo pensare che il dibattito sull'impatto che questo disegno di legge, se approvato, avrà sulle funzioni fondamentali di Province e Comuni non sia una questione fondamentale di cui il Parlamento deve occuparsi. Altrimenti rischiamo di avere non soltanto un regionalismo estremistico e sgangherato che rompe l'unità del Paese, che provoca spostamenti massicci di risorse in direzione sbagliata rispetto a quella che invece servirebbe, ma anche una nuova forma di centralismo regionale che non aiuta in nessun modo a far sì che siamo in grado di corrispondere maggiormente alle attese dei cittadini per quanto riguarda l'erogazione di beni e servizi essenziali.

che si decide di portare nel tessuto vivo di alcuni servizi fondamentali, di alcune fondamentali attività dello Stato. Prevedere che possa essere oggetto di autonomia differenziata la questione delle reti di trasporto, dei porti e degli aeroporti *(Applausi)*; prevedere che possano essere oggetto di autonomia differenziata la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; prevedere che si possa regionalizzare la scuola: ma corrono e di quale rischio all'identità culturale e all'unità nazionale porta la decisione di regionalizzare le norme generali sull'istruzione? tutto questo ci porta a essere convinti che questo provvedimento vada fermato prima ancora che il suo esame inizi. Questo è il significato autentico pregiudiziale e per questo la sosteniamo con molta forza. Abbiamo portato avanti in Commissione una battaglia politica nel merito contro questo provvedimento, una battaglia mirata, portando nella discussione tanti argomenti che purtroppo non hanno trovato l'accoglimento che speravamo. Ultimissima violazione di qualsiasi principio di ragionevolezza - e anche, secondo me, di principi costituzionali - è senz'altro il fatto che noi avremo l'elemento fondamentale di tutto questo processo, e cioè i livelli essenziali delle prestazioni, che non saranno determinati con una legge del Parlamento. gli interventi dei colleghi della maggioranza che diranno che il testo iniziale del disegno di legge prevedeva che i LEP si determinassero per decreto-legge, e siamo arrivati a scrivere che li determiniamo per decreto legislativo. Il decreto legislativo un qualche coinvolgimento del Parlamento nelle Commissioni per il parere lo prevede e, dunque, dovremmo accontentarci. No, noi non ci accontentiamo, perché la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dovrebbe avvenire con un pieno coinvolgimento del Parlamento. Si dice inoltre che, nelle more della definizione degli strumenti con cui si dovrà regolare questa questione, comunque si agirà per decreto e con il peggior decreto possibile in termini di tutela del Parlamento, cioè un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che non ha bisogno - come tutti sapete - ne abbiamo discusso a lungo in altri tempi, di alcuna conversione parlamentare. Quindi, mi pare che i motivi perché questa discussione si interrompa qui, perché la maggioranza faccia una riflessione e perché non venga inferto un colpo così grave all'unità del Paese, una ferita così grande al tessuto istituzionale dell'Italia siano davvero abbondanti. Per questo il Partito Democratico ha presentato la questione pregiudiziale QP4 e poi, in dichiarazione di voto,

Signora Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro subito il voto favorevole del mio Gruppo alla questione pregiudiziale QP1, a prima firma

costituzionali, in particolare agli articoli 1, 3, 4, 33, 34, 53, 70, 116, 117 e 119. Quello in esame è un disegno di legge di riforma che riteniamo scellerato, figlia di una cultura vecchia, perché il provvedimento parte da una cultura di bossiana memoria - come si usa dire - quella in sostanza della secessione.

dare competitività. Si chiama "autonomia differenziata", non autonomia solidale, coesione sociale, riduzione della disuguaglianza. Autonomia differenziata significa Regione competitiva. Quindi, la domanda è come si fa a garantire i LEP, cioè i livelli essenziali di prestazione, se si ritiene di affrontare la questione a costi costanti, e cioè senza oneri per lo Stato rispetto a quelli che si hanno oggi?

fare. Si va invece in direzione di una cultura secessionista e antimeridionalista, perché è la cultura in cui è nata questa proposta. È una cultura antimeridionalista. Io sono del Nord, ho lavorato in fabbrica e ritengo che i lavoratori del Sud abbiano portato una grande cultura e anche

sottointesa sostanzialmente, che i meridionali non hanno voglia di lavorare e che si devono risolvere le cose in casa loro. Questa è la cultura che sta dietro. Attenzione perché all'interno di questa cultura

«È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana». È compito della Repubblica e dei parlamentari rimuovere gli ostacoli, non renderli permanenti. Oggi ci troviamo a vivere un momento che noi speravamo di non dover vivere.

Speravamo che fosse chiaro anche a questa maggioranza e al Governo che parlare oggi di autonomia differenziata è antistorico e anacronistico, perché i divari sono i più grandi di sempre; perché abbiamo più di 5 milioni di persone in povertà assoluta; perché c'è una parte di Paese che non ha accesso ai servizi essenziali. È un progetto antistorico, anche perché nello stesso momento stiamo lavorando per attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha l'obiettivo diametralmente opposto opposto di usare 200 miliardi di euro per rafforzare la coesione territoriale e chiudere i divari. È un progetto antistorico, anche perché la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 ci ha dimostrato che, dando più potere alle Regioni nella gestione di alcune materie, aumentano i divari. Questo non lo affermo io, non lo dice il MoVimento 5 Stelle: lo affermano i dati. Si stima che, da quando è stata fatta la riforma del Titolo V, circa 60 miliardi di euro all'anno vengono sottratti a una parte di Paese; si stima che ci sono 4.000 euro in meno di spesa pubblica che vengono investiti nei cittadini che vivono in alcune Regioni; 4.000 euro in meno spesi in spesa pubblica vuol dire meno sanità pubblica, meno scuola pubblica, meno trasporti pubblici. Questo vuol dire. Personalmente speravo di non dover vivere questa giornata, anche perché al Governo ci sono quelli che si definiscono patrioti, che addirittura hanno l'Italia nel nome del loro partito. Pensavo che i parlamentari che sono seduti qui in Aula, signor Presidente, in realtà rappresentassero tutti quei governatori di centrodestra, quei sindaci di centrodestra che hanno manifestato contrarietà, che addirittura hanno approvato atti regionali e comunali contrari all'autonomia differenziata. Invece eccoci qui, a un anno di Governo, quando evidentemente questa maggioranza ha trovato la quadra e, nell'ambito di uno scambio di potere tra autonomia differenziata, premierato e riforma della giustizia sulla pelle dei cittadini, oggi ci porta a discutere in Aula il disegno di legge Calderoli, che - in questo faccio riferimento a quello che ha detto il relatore

che, permettendo alle Regioni di trattenere il gettito fiscale, sarà minore il gettito fiscale che va nelle casse dello Stato, e non è possibile che non ci sia un profilo finanziario da approfondire. *(Applausi)*. Per questo avevamo chiesto di svolgere un'indagine conoscitiva in Commissione bilancio.

contengono veramente di tutto: dall'energia alla ricerca, dalla scuola alla sanità. Insomma, andremo a creare uno Stato arlecchino con 20 piccole patrie - evidentemente la Lega le vuole - che concorreranno tra di loro per beni

alle Regioni. Il risultato finale sarà quello di cristallizzare le disuguaglianze e le differenze tra cittadini di serie A e cittadini di serie B. Pertanto, quello che oggi vediamo in alcuni ambiti, come per esempio la sanità, diventerà lo stato di fatto anche per tutte le altre materie. Desidero concludere un dato pubblicato su un *report* di ieri uscito sulla stampa. Oggi 9 milioni di cittadini italiani sono in condizione di povertà, anche perché non riescono a sostenere le spese sanitarie, e 4 milioni di cittadini hanno rinunciato alle cure sanitarie. Questo succederà anche per la sicurezza sul lavoro, per i trasporti, per i servizi sociali, per tutte quelle materie da cui deriva il pieno sviluppo della persona umana, come sancisce la Costituzione. Fermatevi, allora, perché siete ancora in tempo. Accettate quello che vi abbiamo detto, quello che magistralmente il senatore Castiello ha esposto, spiegando perché questa legge è anche incostituzionale, e votate con noi a favore

Costituzione, che è il pezzo più importante di quello che noi tutti - qualcuno con un'enfasi che oggi ci sembra esagerata - definisce la nostra Nazione, cioè il luogo dei dei nati, della cultura, della condivisione unitaria di alcuni valori e che fa sì che un bambino che nasce in Italia possa dire di nascere in Italia, di avere dei diritti che siano civili e sociali uguali a quelli di altri bambini su tutto il territorio nazionale.

dal punto di vista definitorio, ma - come si legge nella lettera di dimissioni con la quale i suddetti soggetti si sono dimessi dal Comitato per - anche quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per erogare prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra Stato e autonomia territoriale e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali e - attenzione - quale condizione per l'attribuzione di ulteriori funzioni. Questo comma, che pure è citato anche nella nuova versione della legge, non rispecchia quello che poi c'è scritto nella formulazione della legge, il principio che questa soglia fondamentale, questo nucleo fondamentale che voi avete scritto nella legge di bilancio, e che è citato nell'attuale norma, fa riferimento a un'idea che quelle condizioni devono essere realizzate prima che che si possano erogare altre funzioni. Qui invece c'è un punto che tutti hanno sottolineato, dalla Banca d'Italia all'Ufficio parlamentare di bilancio, ossia l'idea che si possano definire dei LEP, anche laddove la definizione fosse corretta, cioè di livelli essenziali delle prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale, questa definizione deve poi comportare che quei livelli siano effettivamente garantiti. Ebbene, questo presidio, che hanno chiesto la Banca d'Italia e l'Ufficio parlamentare di bilancio - come pure ha ricordato la Commissione europea in un suo commento allo Stato nazionale italiano non c'è da nessuna parte. Anzi c'è addirittura una presa in giro per la quale a un certo punto si passa a decreti legislativi che dovrebbero definire i livelli essenziali delle prestazioni; ma nelle more di quei livelli essenziali delle prestazioni in realtà valgono le definizioni preliminari dei dei livelli essenziali delle prestazioni e comunque quando sono definiti quei livelli, quei livelli sono fatti salvi. Questo allora significa che sostanzialmente già sappiamo - lo hanno commentato economisti e autorevoli giuristi che quei livelli delle prestazioni sono una *fictio*, perché intanto sono basati su una spesa storica e inoltre non esauriscono l'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni che possono e devono essere immaginati. Quindi, partiamo già da un elemento di scarsità e da divari territoriali esistenti. E stiamo andando in un contesto nel quale finiamo per anticiparli e vi è di più: c'è una tensione tra l'articolo 5 e l'articolo 8 della nuova formulazione e anche questo si riflette sotto un profilo costituzionale. Si dice all'articolo 8 che le eventuali relazioni che riguardano le decisioni di compartecipazione fiscale

dopo. Noi stiamo cristallizzando le disuguaglianze e le stiamo aumentando, riducendo le distribuzioni per le altre Regioni, e poi semmai inseguiamo. Quindi, per definizione logica, visto che poi la compensazione è successiva, questo tipo di impostazione crea e alimenta i divari esistenti. È un elemento che va contro la Costituzione e va contro l'articolo 116, che ha una parolina molto importante, che è stata dimenticata - l'ha citata molto bene il collega "inerenti", cioè materie o ambito di materie "inerenti" a ciò che l'articolo 117 dice. Questo elemento è stato completamente superato, per cui la norma che si propone ha carattere carattere dissolutorio. Sostanzialmente si fa una riforma costituzionale nascosta, utilizzando una riforma che peraltro - come è stato molto ben detto - esautora completamente il Parlamento. Se davvero credete di aver fatto una riforma che funziona, perché bisogna esautorare il Parlamento dei suoi poteri e delle sue prerogative? Perché bisogna togliere a questo Parlamento la dignità di rappresentare l'unità del Paese e di rappresentare gli interessi di soggetti che sono diversi? Presidente, in conclusione, vorrei rivolgermi in particolare a quelle forze politiche della maggioranza che hanno il nome "Italia" nella loro denominazione. Mi riferisco alle future "Forza Piemonte", "Forza Lombardia", "Forza Veneto, "Forza Emilia-Romagna"; ai "Fratelli del Piemonte", ai "Fratelli della Lombardia", cioè a quel precipitato che fa sì che quella che spesso viene chiamata Nazione sarà sarà semplicemente un'aggregazione di diversità. Allora io esorto queste forze politiche a rinunciare ad avere "Italia" nel proprio nome, dopo aver condiviso questo disegno di legge che ha evidenti caratteri anticostituzionali. Ritirate il riferimento alla Nazione nei vostri discorsi, alla terra dei nati. Ma anche, vista la non costituzionalità di queste norme, ritirate dai vostri discorsi anche la parola Patria, la terra dei padri, la terra dei nostri Padri costituzionali, che hanno voluto la Costituzione e il Paese unito, libero, solidale.

Oggi noi abbiamo di fronte un disegno di legge che è volto finalmente (dal 2001) ad attuare la Costituzione, ma non solo dal 2001, parlando di questo

Che non sia scritto bene lo si sa; non per niente abbiamo bisogno di questa legge. Abbiamo bisogno di una legge che segni un tracciato, ma un tracciato che oggi è veramente un momento storico. Quello che c'è scritto in Costituzione non è un qualcosa appeso al vento. al vento. Si prevedono dei diritti costituzionali, da dove nasce anche un diritto di noi, delle Regioni, di chiedere quello che c'è scritto nella Costituzione. È un diritto che diventa una pretesa.

Ringraziamo tutta la Commissione e il suo Presidente, ma ringraziamo altresì l'opposizione che porta questi temi, che non fanno che confermare la bontà del percorso dell'autonomia.

paura dei divari, secondo voi attualmente in Italia non ci sono divari e differenze, tutti i cittadini ricevono gli stessi servizi e le stesse prestazioni da parte della pubblica amministrazione. Non è così. Il motivo per il quale noi arriviamo a questo provvedimento è per dare veramente una risposta a quella che è la richiesta del cittadino di avere dei servizi. Che cosa fa oggi la legge Calderoli? Attua un'altra norma fondamentale della Costituzione ancora inattuata, e cioè la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Questa parola, che pochi sanno spiegare e pochi sanno attuare, trova qui finalmente il la per dire che si fanno i livelli essenziali. Ciò significa individuare l'asticella sotto la quale non dovrà essere erogato un servizio; un servizio; l'asticella sotto la quale una pubblica amministrazione non potrà andare nemmeno con i termini di risorse e fa nascere i veri diritti. Ciò per dire che finalmente una legge che prevede regionalismo differenziato potrà dare una risposta

tutte le critiche che sono state rivolte al disegno di legge e devo dire sinceramente che non mi hanno affatto convinto. Mi hanno suscitato invece una domanda

non sono state sollevate quando il Governo di Gentiloni, autorevole esponente del Partito Democratico e Presidente del Consiglio, ha avviato

E allora non c'era nemmeno una legge procedimentale che fissasse le modalità, le condizioni e i termini attraverso cui procedere a queste intese. si dava immediata attuazione al dispositivo della Costituzione, trattando ogni Regione in base ad accordi bilaterali senza regole, all'interno dei quali tali accordi dovevano e potevano essere realizzati. Certo, la legislatura è finita e non siete riusciti a farlo, ma politicamente portate la responsabilità di aver aperto questo procedimento. Noi lo vogliamo fare dando delle regole precise e uguali per tutti. Ciascuna Regione che voglia chiedere la devoluzione di ulteriori materie, ai sensi degli articoli 116 e 117 della Costituzione, lo potrà fare esclusivamente nell'ambito di un procedimento e alle condizioni che noi oggi approviamo. Cari colleghi, non si viola e non si disattende la Costituzione. Si applica la Costituzione. Semplicemente si pongono le condizioni per attuare la Costituzione, che voi avete modificato con soli quattro voti di scarto, alla fine di una legislatura nella quale pensavate, con quella riforma, di agganciare un partito che stava nel campo del centrodestra per portarlo dalla vostra parte: alla faccia di una riforma fatta in nome del popolo italiano, cari colleghi della sinistra! Riforma che poi avete lasciato inattuata per vent'anni, compresa la definizione dei livelli essenziali di prestazione, indicati in Costituzione, da voi ignorati per vent'anni e che noi, invece, grazie alla norma inserita nella legge di bilancio dell'anno scorso, stiamo attuando. Questo perché i cittadini italiani, che risiedano nell'estremo Nord o che risiedano nell'estremo Sud, hanno diritto alle stesse identiche prestazioni e, soltanto attraverso la definizione dei LEP, si può ottenere un tale risultato. E noi abbiamo condizionato il trasferimento di ulteriori funzioni, materie o ambiti di materie alle Regioni che ne dovessero far richiesta al rispetto dei livelli essenziali di prestazione. Caro Presidente, oggi alcuni colleghi si scandalizzano del fatto che che sia possibile, in astratto, trasferire addirittura materie come l'istruzione e l'energia. Ma, collega Parrini, chi l'ha scritta questa norma? L'ha scritta il centrodestra o l'ha scritta il centrosinistra?

cambiare idea sia segno di intelligenza: è vero. Se cambiare idea è segno di intelligenza, allora il Partito Democratico ha certamente il quoziente intellettivo più alto di tutti in avete cambiato idea sul Titolo V. Avete cambiato idea sull'abolizione delle Province. Avete cambiato idea sull'istituzione dei CPR, che voi avete votato. Avete cambiato idea persino sull'abolizione del mercato tutelato, dimenticando che voi l'avete inserito come condizione nel PNRR. Oggi la chiamate tassa Meloni, dimenticando, appunto, che l'avete prevista voi. Avete cambiato idea su tutto: complimenti, siete certamente più intelligenti di noi. Noi ci limitiamo ad attuare la Costituzione. Mi dispiace sentire in quest'Aula che liquidiamo la questione in pochi minuti, otto mesi di discussione, confronto, audizioni, centinaia di votazioni, centinaia di emendamenti esaminati, ottanta emendamenti approvati, di cui oltre la metà dell'opposizione. Se questo voi lo chiamate liquidare l'argomento in pochi minuti, prendo atto che abbiamo una concezione molto diversa del tempo. Questo è, in assoluto, il disegno di legge che ci ha impegnato per più tempo nei lavori in questo inizio di primo primo anno di legislatura. Voi dite che questa legge viola il principio di uguaglianza. Ma, cari colleghi, voi volete dire che i cittadini italiani hanno davvero diritti uguali nel profondo Nord e nel profondo Sud? Ci volete dire che, negli ultimi vent'anni, i divari sono diminuiti, visto che non abbiamo applicato l'autonomia differenziata? Io credo che sia sotto gli occhi di tutti che i divari sono aumentati in questi vent'anni. Attenzione, poi, perché sono aumentati non solo fra Nord e Sud, ma fra centro e periferia, fra zone urbane e zone periferiche, fra montagna, collina e pianura. Attenzione: i divari non sono soltanto sull'asse Nord- Sud, ma sono anche trasversali. Allora, perché negare la possibilità di portare

quel principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione? Altro che violazione dell'articolo 97! Come ci ha bene spiegato il professor Cassese in audizione, noi vogliamo porre le condizioni perché la pubblica amministrazione dia un servizio il più vicino possibile al cittadino.

che in Commissione ha dato un contributo prezioso, che abbiamo accettato e valorizzato, perché ascoltare le critiche è utile anche alla maggioranza, per scrivere meglio le leggi. Nessuno ha la verità in tasca. Abbiamo accettato più di 40 emendamenti dell'opposizione e anche grazie al contributo di Fratelli d'Italia il disegno di legge è stato migliorato. Infatti, abbiamo inserito nell'articolo 1 il principio di coesione nazionale, poi ulteriormente declinato all'articolo 10: altro che spaccare l'Italia! di legge reca all'articolo 1 il principio che l'autonomia differenziata deve avere come finalità il rafforzamento e la realizzazione del principio di coesione nazionale e quindi di uguaglianza tra tutti i cittadini. *(Applausi)*. Abbiamo inserito all'articolo 3, sempre grazie a un emendamento che mi onoro di aver sottoscritto per primo, il principio che si debba passare attraverso il Parlamento con decreto legislativo e non affidarsi ai DPCM, che pure a voi sono molto cari, come la recente cronaca della passata legislatura ci ricorda. *(Applausi)*. Noi abbiamo voluto che si procedesse con decreti legislativi e abbiamo inserito all'articolo 9 il principio di perequazione; abbiamo inserito all'articolo 7 il principio importantissimo della supremazia statale, che vuol dire che lo Stato potrà sempre dichiarare la cessazione dell'intesa conclusa con la Regione, qualora essa sia inadempiente proprio nella salvaguardia dei livelli essenziali di prestazione e dei diritti sociali e civili dei cittadini. Questo abbiamo fatto. Si può migliorare? Certo, ma questo disegno di legge non ha assolutamente la finalità di aumentare il divario fra cittadini di serie A e di serie B, ma ha proprio la finalità di

che domani, quando cominceremo a votare gli emendamenti, ce ne sarà uno, il 4.203, a prima firma De Priamo, che ha già avuto il consenso del Ministro e di tutta la maggioranza, in base al quale anche alle Regioni che non chiederanno la devoluzione di determinate materie

è l'emendamento che propone Fratelli d'Italia e che approva tutto il centrodestra e questa è la ragione per la quale mi sento tranquillamente di poter affermare che le vostre obiezioni sono propaganda politica, che non comprende il significato di questa legge e la ragione per la quale Fratelli d'Italia voterà convintamente contro tutte le pregiudiziali. *(Applausi)*.

del 20 dicembre scorso, in cui ho chiesto al Ministro degli affari esteri informazioni sulla sorte di Ilaria Salis, una nostra connazionale che è reclusa nelle prigioni ungheresi in condizioni che vengono riportate come assolutamente inaccettabili, disumane e degradanti, per un reato francamente risibile. La nostra connazionale è stata accusata di aver aggredito due neonazisti, i quali avrebbero avuto una prognosi di cinque e otto giorni, e per questa ragione è reclusa, con una pena possibile di undici o - si legge - sedici anni di prigione, in una galera nella quale, per intenderci, non ha avuto né vestiti, né assorbenti igienici, né asciugamani. Non è in condizione di mangiare due volte al giorno; viene portata in udienza legata in catene e con una sorta di guinzaglio. Tutto

di rispondere alla mia interrogazione, perché io l'ho scritta il 20 dicembre e la nostra connazionale è ancora lì, a distanza di tre settimane, e rischia di restarci in carcerazione preventiva fino a un anno. Vorrei sapere se sta muovendo le leve della nostra diplomazia per fare in modo che questo governo ungherese dell'Unione europea ci restituisca immediatamente la concittadina Ilaria Salis. Abbiamo visto cosa è stato fatto per Patrick Zaki: quella è la politica. Si opera con il Governo di un altro Paese e si trova una soluzione che magari salvi la faccia a quel Paese, ma si porta indietro il nostro connazionale.

è molto generosa e sono sicuro che la famiglia Salis saprà apprezzare la sua generosità.

ma questo mi è impossibile, perché le interrogazioni parlamentari presentate giacciono da settimane senza risposta e perché il Governo ha deciso apertamente di insabbiare un mio disegno di legge riguardante l'argomento su cui farò alcune brevi considerazioni. L'appello che voglio fare alla Presidente del Consiglio è il cara Giorgia Meloni, si metta una mano sulla coscienza, veramente, e decida di esercitare il potere, che lei ha, di far finire un gigantesco scandalo morale e istituzionale che sta andando in scena in questo Paese. Lo scandalo a cui mi riferisco è il seguente e spero di riuscire a stare nei minuti che mi sono stati assegnati: da mesi il Governo - inopinatamente, devo dire - ha dichiarato guerra ai familiari delle vittime dei crimini nazifascisti nel nostro Paese. A portare avanti questa guerra per conto del Governo e, segnatamente, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze è l'Avvocatura generale dello Stato, che in molti processi usa argomenti assurdi e indegni per difendere la Germania, che è il soggetto citato in giudizio,

e bloccare il pagamento degli indennizzi che sono dovuti soltanto in presenza di sentenze passate in giudicato. Diversamente da quanto sostenuto da una nota di Palazzo Chigi della scorsa settimana, l'Avvocatura generale dello Stato non sta effettuando un doveroso lavoro di verifica della titolarità dei ricorrenti ad essere risarciti. No, sta ponendo in essere un vero e proprio boicottaggio di Stato, perché è vergognoso dire a un ricorrente, figlio perché è vergognoso dire a un ricorrente, figlio della vittima di un eccidio, che non ha diritto al risarcimento perché non era ancora nato quando suo padre fu arrestato per essere deportato in un *lager* dove trovò la morte e quindi non ha sofferto abbastanza. È vergognoso - questo è un altro argomento dell'Avvocatura - dire alle due figlie di uno dei trucidati nella strage di Niccioleta che non devono essere risarcite perché quando avvenne l'assassinio del loro padre erano troppo piccole per soffrire. Ed è vergognoso - ultimo esempio, ma ce ne potrebbero essere molti - parlare di prescrizione del diritto al risarcimento di fronte a crimini così immani, che sono crimini di guerra e contro l'umanità. Vorrei chiedere alla Presidente del Consiglio e anche a tanti Ministri una cosa molto semplice: perché vi comportate così? Che male vi hanno fatto i familiari delle vittime degli eccidi, delle deportazioni e delle stragi di Sant'Anna di Stazzema, di Cavriglia, di Civitella, del Padule di Fucecchio...

e di fare quanto necessario affinché questa vergogna cessi, possibilmente prima del 27 gennaio, quando tutti vorremmo festeggiare unitariamente e a testa alta il Giorno della memoria.

e colleghi, è con un sentimento profondo di tristezza e rispetto che desidero ricordare in quest'Aula la vita straordinaria di Ferruccio Laffi,

della loro casa dalle truppe delle SS. La sua vita, segnata da una ferita profonda, è sempre stata un esempio di resilienza e coraggio. Cinquant'anni di silenzio precedettero la scoperta del cosiddetto armadio delle vergogne, dopo la quale Ferruccio ha dedicato il resto della propria vita a narrare una storia, garantendo che la memoria di quel tragico evento non si perdesse nell'oblio. Nonostante il dolore immenso della perdita insopportabile, Ferruccio ha abbracciato la missione di educare le giovani generazioni, trasmettendo il suo messaggio di tolleranza, pacificazione e amore per la libertà e la democrazia. La sua è stata una vita dedicata all'inno della bontà d'animo, rifiutando di cedere all'odio nonostante la terribile ingiustizia subita. Oggi l'Italia piange la perdita di un eroe, un partigiano riconosciuto dal 1° marzo 1944 fino alla liberazione, un messaggio di pace e democrazia. Ferruccio Laffi ha lasciato un vuoto irrimediabile nel nostro tessuto sociale; la sua capacità di emozionare, la sua dedizione, l'impegno civile e la sua lucida difesa dei valori democratici rimarranno per sempre nella nostra memoria. In questo momento di lutto esprimo le mie più sentite condoglianze, a nome del Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, alla famiglia di Ferruccio Laffi e a tutta la comunità di Marzabotto. La testimonianza rimarrà un faro per le generazioni future, un monito contro l'oblio e un appello costante alla difesa della libertà e della democrazia. Dalla memoria di quel periodo storico, di cui l'umanità ha perso la coscienza e in cui l'indifferenza era l'arma più crudele, gli uomini come Ferruccio sono state delle guide moderne. Grazie, Ferruccio, per il tuo coraggio, la tua intelligenza e il tuo straordinario impegno. Ci mancherai profondamente.

sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

ed altri. -*** ***Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***